interpretare la lettura del processo verbale. Intendo sollecitare nuovamente, come è già stato fatto tante volte in quest'Aula anche durante la scorsa legislatura, la sistemazione dell'impianto di amplificazione. Non abbiamo capito una parola:

Presidente, questa mattina, in chiusura di seduta, il collega Fruscio ha sollevato un problema, che credo sia fondamentale,

chiarisca quanto prima questa questione perché non è assolutamente secondaria e tra l'altro crea un precedente credo pericolosissimo nei confronti delle leggi che regolano la finanza pubblica e delle leggi di bilancio. Sollecito dunque la Presidenza

della legittimità dell'esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita. Non vi è dubbio che questo sia un diritto costituzionalmente garantito, se vi sono delle perplessità sull'opportunità politica dell'esercizio di questo voto nel momento in cui vi è un'Aula divisa in due parti identiche - così come lo è stato il Paese in occasione delle elezioni politiche e dunque un Governo sostenuto dal loro voto, come abbiamo visto anche oggi durante il voto sugli emendamenti. l'opportunità politica che i senatori a vita siano determinanti per la sopravvivenza di un Governo che noi riteniamo estremamente debole, altra cosa è contestare, in maniera errata, secondo me, la loro legittimazione costituzionale. È proprio per questo, anche alla luce delle interessanti parole che abbiamo ascoltato in quest'Aula da parte del presidente emerito Cossiga, che, attraverso la mia dichiarazione, il Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, fa proprio l'Atto Senato n. 681, a prima firma della senatrice Alberti Casellati, che reca: «Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita».

In sostanza, egli ritiene che il contenuto del disegno di legge finanziaria sia contrario alla legge, in particolare perché l'articolo 53 del testo originario modificherebbe, violandole, le leggi di contabilità dello Stato. Nella lettera, il senatore Fruscio ha chiesto anzitutto che il Presidente dichiari irricevibile il disegno di legge finanziaria come approvato e trasmesso dalla Camera. Questo evidentemente è al di fuori dei poteri del Presidente. Quanto ad un diverso intervento del Presidente, va ricordato che i poteri del Presidente del Senato sul contenuto del disegno di legge finanziaria sono diversi in prima e in seconda lettura, secondo il disposto del nostro Regolamento. In prima lettura, il Presidente del Senato accerta se il provvedimento rechi disposizioni estranee al suo oggetto ovvero volte a modificare norme della contabilità generale dello Stato. In tal caso, il Presidente comunica all'Assemblea, se lo ritiene, lo stralcio di queste disposizioni. Sia in prima che in seconda lettura (è il caso che ci riguarda), il Presidente accerta la correttezza della copertura del disegno di legge finanziaria e ne dà comunicazione all'Assemblea. Queste valutazioni del Presidente sono in ogni caso adottate sentito il parere della 5a Commissione e del Governo. È chiaro allora che nella situazione presente, dovendo il Senato esaminare un disegno di legge finanziaria approvato e trasmesso dalla Camera, il Presidente non ha alcun potere di accertare la presenza nel contenuto del provvedimento di norme in materia di contabilità generale dello Stato. Quella sollevata dal senatore Fruscio, è dunque una questione di merito che potrà essere esaminata anzitutto in sede di 5a Commissione. Per questo il Presidente ha informato il presidente Morando dell'iniziativa del senatore Fruscio e della sua risposta.

Presidente, intervengo, come è prassi e consuetudine regolamentare,

Il parere reso, sotto il profilo formale, non presenta inconvenienti, è condivisibile; noi intendiamo porre, invece, alcune questioni fondamentali che riguardano il prospetto di copertura finanziaria e che possono far cadere i propri effetti sulla copertura della legge finanziaria stessa e più ancora, nel corso del tempo, sull'intero rapporto *deficit*-PIL. Due sono le questioni.

è accaduto questo: il Governo aveva introdotto nella legge finanziaria una legge delega. A questa legge delega annetteva copertura per la legge finanziaria di un miliardo di euro. È noto che la legge finanziaria non può contenere una legge delega: il Governo al riguardo ha tenuto un atteggiamento abbastanza inusitato, ma in ogni caso ha espunto dal prospetto di copertura della legge finanziaria il miliardo di euro di euro che annetteva a quella legge delega. In questo modo la finanziaria era scoperta per un miliardo di euro ed il Governo ha pensato di

noi. Nessuno vuole legare i colleghi allo scranno, ma il rispetto di chi sta parlando e anche di chi sta ascoltando dalle tribune mi pare un atto doveroso in assoluto.

Va detto che tra l'importo per la copertura della legge finanziaria e il tetto massimo

di gran lunga superiore a quello necessario per la copertura della finanziaria. Si tratta di un punto politico di grande serietà: a che servono cifre che - ribadisco

Ma la questione politica si pone: come mai in un contesto di difficoltà della finanza pubblica, ci sono questi *spread* che

gli emendamenti, con un evidente peggioramento della finanza pubblica. Nella fattispecie ciò non è accaduto perché il Governo ha ha espunto il miliardo ed utilizzato il saldo prima dell'esame degli emendamenti, ma l'introduzione di questo principio è un fatto molto grave. In tal modo la legge finanziaria si è presentata con un'evidente scopertura cui il Governo ha dovuto sopperire con il ricorso al peggioramento dei saldi. La seconda questione, Presidente, che si pone è la il Governo ha usato un consistente miglioramento del cosiddetto risparmio pubblico a copertura della legge finanziaria. Anche questa non è pratica illegittima, ma perfettamente legittima. Intanto, però, il Governo ha potuto utilizzare ben 7 miliardi di euro per la copertura finanziaria perché aveva disposizione 25 miliardi miglioramento del risparmio pubblico relativo a quest'anno; il che significa che la drammatizzazione fatta dal Ministro del tesoro, in sede di presentazione della finanziaria, era evidentemente pretestuosa e strumentale: egli si è trovato maggiori entrate per 25 miliardi circa

due questioni politiche che in questa sede andavano affrontate e che è necessario siano portate all'attenzione del dibattito pubblico e politico, perché ha significato aver costretto ad uno *stress* fortissimo milioni di cittadini e decine di migliaia di imprese in presenza - ed il Governo lo ha dovuto denunziare in sede di prospetto di copertura - di significative entrate, che sono state usate addirittura a copertura del provvedimento e che, invece, potevano essere usate per ridurre l'aumento delle tasse posto a carico dei cittadini. Questo è il punto politico che volevo sottolineare, ribadendo che il prospetto di copertura di questa finanziaria

del quale abbiamo contestato la effettiva capacità di conseguire gli obiettivi in relazione ad una lotta all'evasione che ha i difetti che abbiamo cercato di denunciare e che continueremo a denunciare; per 7 miliardi di euro, grazie ad un miglioramento del risparmio pubblico. Voglio dire al ministro Padoa-Schioppa che siamo di fronte ad una finanza che certamente rigorosa non è; che quando critica i Ministri precedenti di creatività, sbaglia solo per difetto, perché qui la creatività è davvero tanta e va oltre ogni limite; e, infine, che si avvale di una grandezza significativa di maggiori entrate, alle quali annettete in buona parte valore strutturale e che vengono dalla politica del precedente Governo, una politica di abbassamento di aliquote e di allargamento della base imponibile: il contrario di quella che state facendo con la manovra che stiamo discutendo.

Signor Presidente, nella riunione di poche ore fa delle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato, è svolta un'audizione del vice ministro Intini e del sottosegretario Forcieri che hanno riferito sull'andamento della nostra missione in Libano. Per la verità, non hanno riferito nulla, se non che quella missione non sta facendo nulla.

per le quali la maggioranza dei nostri Gruppi ha appoggiato la missione in Libano, vale a dire il disarmo degli hezbollah, non si Non hanno nulla da fare i nostri militari perché i militari libanesi non chiedono assolutamente nulla perché non stanno procedendo al disarmo.

in modo particolare via terra, il che vorrebbe dire che anche attraverso il territorio siriano possono passare tali rifornimenti.

potrebbe presto avere contro otto Ministri, che lo costringerebbero alle dimissioni, tutti questi elementi ci portano a

che rimangono integre rispetto alle considerazioni fatte questa mattina e rispetto alle quali non mi sembra che possa definirsi esaustiva

della facoltà di introdurre in questo momento il testo della legge finanziaria, perché ci sono problemi a monte che non può sottacere a quest'Aula. Scusi, signor Presidente, è vero che può fare ciò che ritiene e ciò di cui si assume evidentemente le responsabilità, ma io sono qui a dirle: perché? Perché non declinare all'Aula la scelta di riflettere su fattispecie che sono di moralità politica, di costituzionalità, di legittimità, di legalità? È vero che il Regolamento sta dalla sua parte, ma perché non deve fare uno sforzo? *(Applausi

Presidente, sarò brevissimo. Intendo far riferimento all'intervento del senatore Selva.

abbiano immaginato di scendere in piazza crea le condizioni per una possibile guerra civile: ci sono quindi tutte le condizioni perché si determini grande preoccupazione. Signor Presidente,

al Governo che venga qui a presentare e a proporre iniziative di natura politica, perché l'impegno delle nostre truppe coinvolge il nostro Paese in termini quanto mai impegnativi. Signor Presidente,

Sulla rilevanza della questione che ha posto e sul fatto che si tratti di una situazione che si aggrava da un giorno all'altro, non mi sento di obiettare. Ciò che posso fare,

grazie ad un impegno continuo dei deputati della Lega Nord che negli ultimi anni hanno ripetutamente presentato pochi emendamenti e proposte a favore dei cittadini e delle imprese del Piemonte colpiti dall'alluvione straordinaria e distruttiva del 1994, è stato consentito anche ai soggetti colpiti dall'alluvione del novembre 1994 di definire, in via automatica, la propria posizione tributaria, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, analogamente a quanto già previsto dalle scorse leggi finanziarie per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. Tali agevolazioni tributarie, insieme al decreto ministeriale che permette la rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate secondo i danni effettivamente subiti, hanno dato nuove possibilità alle nostre imprese piemontesi, tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche distrutte dalle alluvioni. Il presente emendamento propone una proroga del termine per la presentazione delle domande per venire incontro alle difficoltà riscontrate dai contribuenti a causa della mancata informazione.

diceva che i lavoratori e i pensionati non arrivavano a pagare il latte e il pane a fine mese. Vorrei ricordare che l'aumento del gasolio non lo ha stabilito il Governo Berlusconi, ma lo sta facendo questo Governo delle tasse. Si tratta di un aumento che andrà a colpire soprattutto i poveri, perché in macchina, cari amici della maggioranza, non ci vanno solo i ricchi, ma tutte le persone,

la pubblica amministrazione - sto facendo riferimento alla discussione della cosiddetta riforma Frattini - è una risorsa per il Paese, ma lo è a due condizioni politiche, grande professionalità, ma anche grande autonomia. Guai a ipotizzare nella figura della dirigenza un rapporto di scambio, di sottomissione, al cosiddetto potere politico. Così parlava l'onorevole Bressa, e poi... Voi asservite, in maniera grave, la dirigenza pubblica alla volontà della politica e, oltretutto, avete congegnato alcuni meccanismi, tendendo a organizzare un modello cubano - che per voi potrebbe rappresentare un vanto, ma non in cui la burocratizzazione e l'ossequienza al *líder máximo* diventano il paradigma di riferimento continuo delle vostre azioni legislative. Questo *boomerang* ve lo rimandiamo perché con questo provvedimento voi mandate a casa tutti i dirigenti e tutte le possibili dirigenze che non sono state di vostro gradimento, non solo con la riforma Frattini. In più, dite anche che a queste persone, che mandate a casa perché sospettate di avere in qualche modo colluso con il centro‑destra, pagate lo stipendio fino al 2009. Questo è il vostro risanamento. *(Applausi

2.34 propone l'estensione al settore della pesca marittima dei benefici degli agricoltori in materia d'IVA.

dispari di competitività rispetto a nuovi grandi Paesi emergenti sulla scena mondiale. In pratica, signor Presidente, gli agricoltori italiani oggi hanno una redditività molto più modesta rispetto al passato

ma darebbe un ristoro estremamente utile all'intera platea degli agricoltori italiani, ben distribuiti nei vari settori politici rappresentati in questo emiciclo.

uno sviluppo industriale elevatissimo, ma che hanno comportato, però, anche gravissimi danni di tipo ambientale. Ciò anche in ragione di una programmazione economica nazionale - ai tempi in cui questo era oggetto e responsabilità del Governo centrale che, per esempio, ha destinato alla mia Regione il ruolo di grande piattaforma di raffinazione, attraverso gli impianti della chimica di base, fortemente inquinanti, che hanno prodotto un rapporto bassissimo tra capitale investito

con una percentuale di 500 nati sugli ultimi 10.000 nel territorio di Gela, secondo un rapporto di causalità assolutamente accertato tra gli impianti di raffinazione e tali esiti neonatali. è il diritto ad un ecoindennizzo (per così dire, in termini giuridici), ad un giusto risarcimento per tale gravissimo danno, che ha consentito al resto del Paese di godere di un'opportunità sul piano della politica industriale.

durante la discussione della legge finanziaria, di aumentare la quota di spettanza regionale sulle accise per i prodotti petroliferi, spostandone una quota importante dallo Stato centrale alla Regione; di favorire un programma strutturale di recupero ambientale di quei siti; e, infine, di finanziare un grande programma infrastrutturale dei territori regionali aggrediti da tali interventi, per colmare quel drammatico *gap* che separa le Regioni meridionali dal resto del Paese e che, ancora oggi, è condizione

delle autonomie locali - favorisca il recupero ambientale ed un grande programma infrastrutturale, compensando la disattenzione, fino ad oggi elevatissima, che il Governo centrale ha riservato ai territori meridionali.

contiene una puntualizzazione rispetto agli emendamenti illustrati dal collega senatore Pistorio perché riguarda un intervento che si ritiene di dover attuare per un riequilibrio dei tributi afferenti la Regione siciliana. Normalmente - forse in modo troppo facile - viene utilizzata rispetto ai tributi l'argomentazione per cui quelli di essi che si formano in una Regione a Statuto speciale, e quindi in special modo per l'argomento che sto trattando nella Regione siciliana, appartengono alla Regione. Dove si fonda questo assunto? Sappiamo che fonte principale di diritto e quindi il riferimento per la formazione legislativa nelle Regioni a Statuto speciale, quindi nella Regione siciliana, è lo Statuto della Regione siciliana. Per l'appunto, in tale Statuto viene detto che i tributi che si pagano in Sicilia sono della Sicilia stessa, ma questa affermazione rimanda poi la quantificazione alle norme di attuazione. Cosa succede e qual è la diversità della Regione siciliana rispetto alle altre Regioni a Statuto speciale? Mentre per quanto attiene all'IRPEF, quindi all'imposta sulle persone fisiche e all'IRPEG, la quota stabilita come afferente al tesoro siciliano è di dieci decimi, diversamente viene fatto in altre Regioni; ad esempio, in Sardegna, dove la quota è di sette decimi. Tuttavia, questa parte viene compensata in modo squilibrato dall'imposta di fabbricazione. Quando si fece questa norma di attuazione, non si pensava che tale imposta di fabbricazione dovesse essere così rilevante e si riteneva, comunque, che dovesse esserci un contributo per il mantenimento di funzioni nazionali e per il raggiungimento di obiettivi in campo nazionale, quindi la pubblica istruzione secondaria, la difesa e l'ordine pubblico. Di fatto, questo 2 per cento, per la particolarità della Regione siciliana, cioè per il fatto che circa il 50 per cento della trasformazione degli oli minerali avviene in Sicilia, è diventata una cifra molto, ma molto rilevante. Di contro, che cosa è successo? Negli anni, in ultimo quest'anno e precedentemente nel 1996, la quota relativa alla contribuzione della Regione siciliana per le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in Sicilia, e quindi la quota di contribuzione al servizio sanitario nazionale, è stata aumentata per la Regione siciliana e diminuita per lo Stato. Ciò è accaduto l'ultima volta nel 1996, con il Governo Prodi e il ministro Bindi, oggi

una conseguenza rispetto alla spesa che la Regione siciliana deve effettuare nelle zone per mantenere i livelli essenziali di assistenza, chiediamo una parte di questa imposta di fabbricazione che è diventata rilevante. Non è diventata proporzionale con quello che era il motivo per cui, nelle nelle norme di attuazione, veniva stabilito, per il mantenimento delle funzioni nazionali e per il raggiungimento di obiettivi nazionali, la partecipazione dei tributi che venivano ad essere formati nella Regione siciliana. Questo è diventato un motivo di grande interesse ed è l'unico modo per riequilibrare quella che è una contribuzione che diversamente sarebbe assolutamente sproporzionata.

si riferisce ai tassi ipotecari ed è finalizzato a proporre una tariffa più equa di quella prevista nella formulazione dei commi 65 e 66 del provvedimento al nostro esame.

tariffa da 0,516 agli attuali 0,70 euro per ogni soggetto, a fronte dell'aumento del ben 470 per cento dell'attuale costo degli elenchi dei soggetti forniti dall'Agenzia del territorio utilizzati da aziende specializzate per l'erogazione di servizi di monitoraggio ipotecario. Tale aumento è riferito ad un nuovo servizio di trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti oggi non ancora disponibile, come è stato specificato in una

e completa. Appare evidente, quindi, come la disposizione del decreto-legge preveda un passaggio graduale a regime di nuova introduzione. Non trova, quindi, alcuna giustificazione un aumento di tale portata dell'attuale tariffa nelle more dell'attivazione del relativo servizio telematico, dal momento che l'elenco continua ad essere fornito ai richiedenti su supporto cartaceo. Voglio sottolineare

Signor Presidente, intervengo per illustrare i motivi per i quali tutti i Capigruppo di minoranza rappresentati in quest'Aula hanno

Quindi, se anche il Parlamento dovesse abrogarle, accogliendo la nostra proposta, non vi sarebbero riflessi e ricadute, quanto a maggiori spese-minori entrate. Ciò che ci interessa sottolineare in questa sede è l'aspetto di mostruosità giuridica contenuta nel provvedimento al nostro esame, che il ministro Di Pietro, dando l'evidenza di un grande spessore culturale e giuridico, ha inteso imporre con un atto di arroganza nei confronti dell'intero Governo. Signor Presidente, si tratta di una norma con la quale il Governo rinnega atti da sé stesso sottoscritti liberamente e bilateralmente, atti concessori nei confronti di società private, alcune delle quali quotate in borsa, atti che hanno visto riconoscersi la legittimità formale in una riunione del CIPE nel 1997, presieduta dall'attuale presidente del Consiglio, professor Romano Prodi.

nella volontà dell'Esecutivo di bloccare le opere infrastrutturali nel nostro Paese, di rinnegare tutto ciò che era stato avviato nella precedente legislatura dal Governo Berlusconi in termini di maggiore attenzione alla realizzazione di nuove strutture), è una questione giuridica dirimente, signor Presidente. Può un Parlamento libero, democraticamente eletto, suffragare un atto di arroganza di un Ministro il quale un bel giorno stabilisce e dichiara, con un decreto che ha carattere di urgenza, di rinnegare tutti i patti sottoscritti anni fa, patti in virtù dei quali società private hanno ritenuto di indebitarsi sui mercati internazionali, hanno organizzato i loro piani finanziari, hanno individuato un *break-even* in ordine al quale hanno gestito in questi anni le opere pubbliche? Può un Ministro fare queste cose senza che il Parlamento recuperi un minimo di dignità *(Applausi

hanno *extra* profitti esagerati, perché in questi anni hanno guadagnato più di quello che prevedevano i piani finanziari sottoscritti nel 1997, la strada c'era. Bastava applicare un articolo delle convenzioni, rimettere in discussione i piani finanziari, obbligare queste società a ragionare con il Governo e con i rappresentanti dell'ANAS,

siamo stati confortati da tante persone di buonsenso. Una di queste è il magistrato del tribunale di Genova, Michele Marchesiello, che conosco da anni.

questa procedura, sottolineando, nel dispositivo con il quale ha trasmesso gli atti a Bruxelles, che vi sono vari punti critici: aver consentito all'ente ANAS di surrogarsi alle società private e immaginare di intervenire, come si è fatto,

Si tratta di una norma che consente di effettuare i dragaggi nei porti del nostro Paese. Il presidente Prodi e il vice ministro De Piccoli stanno sottolineando da tempo un grande interesse per la portualità italiana. Anche noi riconosciamo che la portualità italiana è alla vigilia di una grande fase di crescita. Infatti, se è vero che la Cina, l'India e il Giappone sono destinati a diventare il centro del mondo (l'istituto Einaudi ha calcolato che nel 2010 in quei Paesi si produrrà il 55 per cento della ricchezza mondiale), è ovvio che in Cina e India (e soprattutto in Cina, finché durerà il regime comunista militare) non ci saranno mercati di consumo e quindi i cinesi saranno costretti ad esportare.

l'occasione storica di calamitare la globalizzazione di ritorno, di fare dei porti, della logistica, dei retroporti un fattore di ricchezza importante. C'è però un piccolo particolare: un centro di studi e di ricerca ha calcolato che in questo momento nel mondo si stanno costruendo 1.100 navi, ma il 60 per cento di esse non potranno mai attraccare nei porti italiani, finché nei porti italiani non si faranno le attività di dragaggio necessarie. In Europa si fanno i dragaggi, in Italia no, perché purtroppo in un Paese che dispone di un pacchetto di leggi superiore a 100.000 non c'è ancora una legge che riguarda e regolamenta i dragaggi.

cosa stabilisce il comma 143? Stabilisce il declassamento a decreto ministeriale degli statuti degli enti di ricerca italiani non strumentali afferenti al Ministero dell'università e della ricerca. una manovra che non ha eguale in tutto il mondo occidentale, nemmeno la Romania di Ceausescu ha messo in questo modo il piede sopra la ricerca. Mi domando come si sia potuti addivenire ad un manovra di questo genere, che è veramente e gravemente lesiva del prestigio della nostra ricerca.

alle usuali verifiche in Commissione bicamerale. Approfitto dell'opportunità di parlare, signor Presidente, per un altro breve commento. Il provvedimento alla nostra attenzione

oneri su oneri, una «selva selvaggia» di imposizioni fiscali. Ne voglio citare alcune: al comma 71 viene modificato il regolamento riguardante le auto promiscue. Ci sono 410.000 italiani che usufruiscono, come dipendenti, di un'auto promiscua: questi signori si vedranno tassato un reddito derivante dall' utilizzo dell'auto promiscua in termini maggiori rispetto al passato per un ammontare di 600-700 euro l'anno, quando mediamente hanno 60.000-70.000 euro l'anno di retribuzione lorda.

Questi, da decine e decine di anni, utilizzano la loro auto potendo dedurre i costi al 50 per cento. Questa norma glieli fa dedurre al 25 non solo lo fa a partire dal primo gennaio 2007 ma per l'anno di imposta in corso. Vi rendete conto in che modo procediamo? Altro che statuto dei contribuenti! È un fatto molto grave. Pensate agli oneri che i professionisti italiani di colpo si troveranno sul loro bilancio di quest'anno.

29, che modifica la tassazione agevolata delle *stock option*, stabilita solo qualche mese fa dal decreto Bersani-Visco (legge n. 223). A parte il dilettantismo legislativo di fare e poi disfare, a distanza di pochissimi mesi, comunque la norma attuale che adesso ci apprestiamo a votare risulta notevolmente più severa di qualunque altra norma sulle *stock* *option* esistente in Europa. risultato è che avremo un impedimento, perché questo è uno strumento formidabile per l'innovazione, per la crescita e per lo sviluppo. Le *stock* *option* sono infatti uno strumento di incentivazione allo sviluppo. lo abbiamo dimenticato e anche per questo avremo una limitazione alla nostra competitività.

acquisiti mediante contratti di locazione e finanziaria, contratti di *leasing*, l'indeducibilità del canone di *leasing* relativo alla quota di capitale imputabile ai terreni pertinenziali. In spregio alla legge dello Stato denominata Statuto del contribuente, questa indeducibilità si applica per i contratti di *leasing* già stipulati e al periodo di imposta in corso. In questo modo, si aggrava di colpo il costo di uno strumento finanziario importante per l'imprenditore e, ripeto, non si tratta di poca cosa: stiamo parlando di 1,5 miliardi all'anno. È uno dei capisaldi dell'entrata vera di questa manovra perché, come ha detto questa mattina, sottolineando bene la composizione della manovra, il senatore Azzollini, per quanto riguarda i risultati della lotta all'evasione e all'elusione, si tratta di una promozione dell'accertamento ma di una scarsissima (uno a dieci) promozione dell'incasso.

emendamento ha lo scopo di abrogare i commi dedicati ad una estensione del sistema delle spoglie, perché questi commi prevedono addirittura due misure *contra personam,* rivolte cioè verso due identificati direttori di agenzia, così come si vuole porre fine, secondo criteri discrezionali, a rapporti di lavoro, di diritto privato che riguardano dirigenti di seconda fascia che non appartengono alle amministrazioni pubbliche. Segnalo a questo riguardo il problema che potrà e dovrà, a mio avviso, porsi a proposito della responsabilità contabile, che potrà cioè derivare nei confronti di coloro che decideranno di porre fine a questi rapporti con gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di diritto privato. Credo però che, soprattutto dal punto di vista politico, sia grave la volontà di produrre uno *spoils system* generalizzato e riferito anche alla dirigenza di seconda fascia. In questo modo si minano la neutralità, l'imparzialità, l'orientamento al risultato, che vengono invocati per le funzioni dirigenziali; in questo modo si vogliono produrre funzioni asservite alla funzione politica.

riguardano quella parte del decreto che istituisce una Agenzia di valutazione dell'università e della ricerca, e 2.166, che riguarda i poteri che il decreto dà al Governo per il riordino degli enti di ricerca.

con quanto prescritto dai commi 138 e seguenti del decreto qui in discussione, vediamo che i compiti della nuova Agenzia sono identici a quelli dei due istituti già esistenti. Non vi è nemmeno una chiara distinzione rispetto a quanto già previsto nella cosiddetta legge Moratti, il decreto-legge n. 7 del 2005, non vi è proprio nulla di nuovo. Di nuovo c'è solo l'accorpamento dei due enti attuali. Dirò subito che non ci è piaciuto il metodo e la vaghezza di contenuti con cui è stato realizzato questo accorpamento. Anziché farlo con un provvedimento *ad hoc*, su cui avviare un serio dibattito parlamentare, si è usato lo strumento di un decreto fiscale. Non comprendiamo le ragioni di tanta fretta. Si dice, per giustificare questo provvedimento all'interno di un decreto‑legge, che sarebbe necessario stabilire la terzietà di una agenzia di valutazione. Il punto è che di questa terzietà qui non vi è alcuna traccia.

Stupisce, al proposito, che nel decreto non si dica chi comporrà l'ANVUR, né, soprattutto, da chi saranno nominati i suoi componenti. Si dà una delega generica e molto ampia al Governo senza nemmeno definire i limiti di durata degli organi direttivi di siffatta agenzia. Tutto questo non è secondario, dato che, quanto già stabilito dalla legge Moratti, il giudizio dell'ANVUR fornirà il criterio per allocare le risorse a università ed enti.

e qui voglio ricordare che proprio la maggioranza ha dato invece atto all'*ex* ministro di aver rispettato criteri non politici, sostanzialmente imparziali nella composizione dei due istituti esistenti. Circola il nome di Berlinguer come futuro presidente: se fosse vero si capirebbe il motivo di tanta fretta! Di estrema gravità, non esito a definirlo eversivo dell'ordinamento costituzionale, è poi il contenuto dei commi 143 e seguenti. Si attribuisce ad un semplice regolamento ministeriale il potere di determinare lo scorporo di strutture degli enti di ricerca, accorpamenti, fusioni, soppressioni. Con un semplice regolamento potremo avere la soppressione e la disarticolazione del CNR, senza che il Parlamento possa impedirlo. È una grave violazione dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione, che stabilisce il diritto per gli istituti di alta cultura di darsi ordinamenti

dell'energia. La 7a Commissione, su iniziativa di Alleanza Nazionale, ha dichiarato all'unanimità «inopportuno» procedere con regolamento al riordino degli enti: siate ora coerenti! Il vero scopo di questo provvedimento appare uno solo: quello di mettere le mani sulla ricerca italiana!

e la serietà della nostra ricerca, di non votare questa norma aberrante. Noi oggi, in Aula, diamo voce allo sbigottimento, al timore e alla indignazione della ricerca italiana.

Chiediamo la possibilità di condividere anche le linee di adozione dei produttori secondari, oltre che, ovviamente, le linee della rete principale. Si tratta semplicemente di dare ad un produttore secondario la condivisione degli impianti esistenti.

con la quale abbiamo cercato di far capire, oltre all'aspetto di costituzionalità ed illegittimità delle norme contenute nei ricordati commi dal 159 al comma 162, anche l'aspetto più odioso di questo provvedimento che riguarda lo *spoils system* violento. *spoils system* è stato inventato dalla legislazione Bassanini ed ha creato un clamore incredibile nel nostro Paese.

disfacendosene, senza capire la grande professionalità acquisita con gli investimenti che lo Stato ha fatto. Ebbene, spero che saranno accolti gli emendamenti soppressivi dei commi ricordati.

facciamo questo ragionamento. Considerati i risultati non positivi che il meccanismo dello *spoils* *system* ha avuto nelle gestioni dei Governi di centro-sinistra e di centro-destra, eliminiamolo completamente. Ritorniamo a far sì che la disciplina della dirigenza dello Stato e degli enti amministrativi dello Stato sia rimessa al diritto pubblico.

della difesa, lo stesso ordinamento di diritto pubblico viene esteso a tutti gli altri dirigenti dello Stato, soprattutto della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Con questo emendamento cerchiamo di dare un un taglio anche a leggi che abbiamo fatto noi; blocchiamo tutto e diamo serenità, importanza e riconoscimento delle professionalità alla dirigenza dello Stato, che oggi risulta impaurita e mortificata. mortificata. L'ho detto in Commissione e lo ripeto qui: ogni Governo ha bisogno della pubblica amministrazione; la pubblica amministrazione e la dirigenza sono la garanzia e la tutela della democraticità del nostro Paese di fronte al mutare delle alleanze di Governo e dei Governi.

Grazie

soppressi, così come chiesto dagli emendamenti dei colleghi Possa e Valditara. Quei commi autorizzano il Governo, con regolamento, al riordino degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università, ma non indicano gli enti da sottoporre alla cosiddetta declassificazione.

Colonnetti. Ora, Presidente, il motivo per il quale era stata prevista una tutela costituzionale per questi enti, attraverso l'articolo 43, è molto chiaro:

di quella che si era verificata nella Romania di Ceausescu *(Applausi dal Gruppo FI)*, dove il problema fu risolto attraverso l'assegnazione della presidenza dell'ente alla moglie, piuttosto che attraverso una degradazione come quella alla quale stiamo assistendo. Il secondo aspetto concerne

ma se questo dovesse essere degradato si verrebbe a trovare in una situazione sott'ordinata rispetto a enti molto meno importanti (cito solamente il CRA e l'ENEA). Per

Lo stesso parere della settima 7a Commissione va coraggiosamente in questo senso. Allora, il mantenere questa disposizione può voler dire due cose:

Presidente mi scusi, ma a pensar male qualche volta si coglie nel segno; sarebbe come sparare con i *bazooka* ad un passerotto.

Non solo credo di dover dire che stiamo correndo il rischio di mettere in gioco il prestigio internazionale del nostro Paese, ma soprattutto vorrei ringraziare alcuni colleghi

In effetti, Presidente, dobbiamo lamentarci, sottolineare e stigmatizzare il fatto che i relatori non stanno dando, come da prassi, da uso, da rapporto di collaborazione e dialettica, da confronto tra le parti, nessuna soddisfazione alla nostra illustrazione. Quindi, la loro contrarietà non viene giustificata né tecnicamente, né politicamente, per quanto la tecnica possa essere distinta dalla politica e la politica dalla tecnica in quest'Aula. C'è di più:

il fatto che il Governo e i relatori non diano nessuna giustificazione alla loro pronuncia non possiamo che intenderlo come un volersi sottrarre a un rapporto di collaborazione

abbiamo ridotto all'osso gli emendamenti e, oggettivamente, siamo quasi arrivati alla fine e stiamo per votare e non c'era neanche bisogno di scomodare auguste figure della Repubblica per farle venire a votare, perché la maggioranza ha retto.

senza prenderci in giro. Credo che l'opposizione abbia il diritto di manifestare indignazione per l'insensibilità dimostrata nei confronti degli

Signor Presidente, l'emendamento 2.1000 prevede che in conseguenza alle minori entrate correnti del bilancio dello Stato, con l'esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente dalla legge, si possa corrispondere con risparmi che tengano conto del delta derivato dalle minori entrate stesse, in tutta coerenza con la necessità di dare a questo decreto una validità sostanziale di equilibrio. Si tratta di una soppressione ampia e dalla portata culturale. Dal decreto-legge sono previste maggiori entrate per 6,6 miliardi di euro dei quali oltre 4 ascrivibili alla lotta all'evasione, principio che noi condividiamo all'interno di una politica fiscale di costruzione di un Paese più moderno e giusto proiettato verso la competitività. Il modello proposto in questo decreto, però, è criticabile perché pervaso da varie iniziative, spesso non coordinate, che non supereranno un endemico male culturale

Dichiaro aperta la votazione.

Dichiaro aperta la votazione.

Signor Presidente, con questo emendamento si tenta di correggere un errore, perché la condizione della quotazione per le *stock options* non va verificata al momento dell'attribuzione dell'opzione, ma al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'assegnazione delle azioni sottostanti. Certo avremmo preferito la presenza in Aula del ministro Padoa-Schioppa per verificare questa situazione, ma troviamo singolare l'indifferenza del Ministro nel seguire l'andamento dei nostri lavori.

questo emendamento riguarda la perequazione tra pescatori e agricoltori ai fini dell'IVA. Si tratta di colmare una disparità di trattamento che non è assolutamente funzionale ad un migliore esercizio della pesca, che particolarmente gravata dalla riforma della pesca mediterranea approvata proprio nella giornata di ieri a Bruxelles e che danneggia fortemente i nostri pescatori. Ricordo ai colleghi del centro-sinistra

Prego, senatore Strano.

saranno comunque ulteriori ricorsi, visti i valori di inerenza che sono stati scritti e che sono assolutamente ingiustificati: è ingiustificato cioè il livello

ci ritroveremo con una nuova sentenza della Corte di giustizia europea che condannerà lo Stato italiano a rifondere le imprese delle somme che, nei prossimi anni, non potranno

Dichiaro aperta la votazione. *(Segue

Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che prevede l'introduzione di un imposta sostitutiva, una cedolare secca per gli affitti. Si tratta di uno strumento importante per combattere l'evasione in questo campo e

stante l'orientamento di voto contrario su tutti gli emendamenti per difendere il testo così com'è, voteremo contro l'emendamento 2.47, ma ne apprezziamo lo spirito e la sostanza e ci proponiamo, come abbiamo detto anche nel corso della discussione

una nostra battaglia, alla quale, concordemente a quanto espresso, vorremmo aggiungere la detraibilità, quanto meno parziale, da parte di colui che

Presidente, con questo emendamento l'UDC ha posto due questioni irrisolte in questo decreto.

Avete pensato o immaginato di dare soluzione con una formulazione ambigua, che troveremo poi negli ordini del giorno; vorrei già dire fin d'ora che cosa stavate immaginando quando avete presentato un primo ordine del giorno, forse pensavate ai PACS.

che non può essere identica a quella per le successioni familiari. Noi dobbiamo favorire i passaggi generazionali

ed una superficie americana media di 500 ettari. Mi rivolgo, in particolare, alla senatrice Thaler della SVP come pure tanti altri amici che trovo dall'altra parte: un coltivatore diretto della provincia di Bolzano, con due ettari di terreno, verrà gravato dell'imposta di successione. Pensiamoci*.

**Il Senato non approva.**

proponiamo, in maniera assolutamente coerente con le norme di contabilità, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. È una questione di grande rilievo. La maggioranza attuale ha affermato più volte in campagna elettorale che avrebbe potuto farlo. Gliene stiamo dando l'occasione; spero la colga, altrimenti gli italiani capiranno. [FRANCO

L'eliminazione dell'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale era un punto qualificante del programma delle Casa delle Libertà, come d'altra parte, nel

potrebbe passarvi per l'anticamera del cervello ammetterlo e ritenere che il ritorno al voto dei cittadini nella prossima primavera sia l'unica soluzione per mostrare chi in campagna elettorale ha detto detto cose serie e puntuali e chi, invece, a distanza di pochi mesi, ha dimostrato di aver mentito sotto uno dei profili più importanti (ce ne sono anche altri: guerra in Libano, eccetera), quello che che avete usato nei confronti dei cittadini come strumento per ottenere consenso elettorale, sapendo già dall'inizio che non avreste rispettato il patto da voi sottoscritto. Il voto favorevole

Avete dimenticato di allineare la deducibilità, oltre alle attività di lavoro autonomo anche per le imprese, pensando che tutte le imprese ne facciano un uso differente rispetto a quello per la finalità d'impresa. Fate in modo che vi sia la procedura di interpello, così che possa essere affrontata attraverso misure antielusive particolari, ma non procedete in maniera indiscriminata, facendo saltare i conti delle imprese. Grazie, senatore

Signor Presidente, questo emendamento è importante perché riguarda l'introduzione della convenzione unica, che pone seri e irrisolti problemi giuridici.

in modo autoritativo e unilaterale una modificazione del rapporto di concessione tra ANAS e società concessionarie. Bisogna notare bene che i concessionari sono stati individuati con gara pubblica e sono società quotate in Borsa che hanno azionisti risparmiatori: non sono ricchi che piangono, ma anche risparmiatori dei fondi comuni. soggetti hanno investito sulla base di uno Stato di diritto dove le regole non si cambiano durante il gioco. Chi non accetta le condizioni del ministro Di Pietro fa i bagagli: questo è scritto nella norma. chi non dichiara di aderire alla convenzione unica decade automaticamente dalla convenzione. E cosa succede se interviene la decadenza automatica? Subentra l'ANAS in una gestione provvisoria. Ma l'ANAS non è una società per azioni? Viene così ripubblicizzata?

Come può subentrare un soggetto privato individuato con gara ad un altro soggetto privato individuato, invece, senza gara? Chi pagherà le spese di gestione nella fase successiva alla decadenza? La gestione della rete autostradale, nel momento in cui viene presa in carico dall'ANAS, dev'essere pagata e la norma non individua nessuna copertura finanza, non è previsto

Il sistema di norme riguardanti la convenzione unica va contro princìpi elementari di Stato di diritto, di civiltà giuridica, di diritto comunitario, come qui è stato ricordato. Siamo a favore della soppressione L'UDC vi rivolge un invito, amici del centro-sinistra, sempre più stretti e vincolati, non solo da componenti politiche radicali, ma anche da componenti politiche che fanno giustizia sommaria perché nella loro vita hanno fatto giustizia sommaria e vogliono fare giustizia sommaria anche della civiltà giuridica di questo Paese. *(Applausi dai Fermateli, finché siete in tempo! E mi rivolgo alle coscienze più libere e democratiche del centro‑sinistra.

chi ha compiuto la valutazione di compatibilità comunitaria di questa norma? È stato forse il ministro Bonino? La stima che nutro per il ministro Bonino mi impedisce di credere che abbia dato il suo assenso ad una norma chiaramente in violazione quella comunitaria e tale da esporci al ludibrio in sede comunitaria. Questo Governo, che era solito rimproverare a quello precedente la mancanza di spirito comunitario, sta percorrendo un cammino lungo il quale incontriamo il massimo di conflittualità

Noi abbiamo molto apprezzato che la maggioranza non abbia posto la questione di fiducia. Chiediamo la soppressione di quest'emendamento. Nel caso venga accolta la nostra richiesta, la manovra finanziaria non subirà alterazioni,

Presidente, lei sa quanto io la rispetti, però vorrei chiederle di cronometrare il minuto che mi spetta, perché nell'intervento precedente ho avuto chiara la sensazione che lei non mi abbia fatto parlare per un minuto. Mi perdoni,

in quell'occasione, il presidente Romano Prodi si è vantato di aver varato la norma sui dragaggi; il ministro di Pietro, con enfasi, ha affermato: «L'ho imposta io!»; il ministro Bianchi ha esclamato: «È la volta buona, io l'ho avallata!». È stato sufficiente che il ministro Pecoraro Scanio facesse uno starnuto

perché altrimenti i porti italiani moriranno di asfissia, le grandi navi, i porta-*container* che transiteranno dalla Cina via Suez in Italia non potranno attraccare e quindi perderemo i vantaggi della globalizzazione di ritorno. Quindi, queste poesie che Romano Prodi fa sul futuro dei porti si areneranno dentro i porti non dragati.

contro l'emendamento 2.101 e informare i colleghi di un fatto molto importante. È vero che su richiesta dei Verdi - e non solo di essi - tale testo è stato stralciato da questo provvedimento, ma subito dopo abbiamo provveduto a convocare un tavolo interministeriale, Trasporti, Ambiente e Infrastrutture...

ha già trovato una soluzione concordata che consente di dragare nei porti, al contempo bonificando e salvando l'ambiente, perché non è soltanto un interesse del centro‑destra far sì che il nostro sistema portuale sia più competitivo rispetto al sistema attuale.

l'emendamento 2.105 riguarda il ponte sullo Stretto di Messina. Colleghi del centro-sinistra, sulla Sicilia fermatevi! Il 2 dicembre terremo, come UDC, una manifestazione nazionale a Palermo per testimoniare la solidarietà e l'amicizia degli italiani ai siciliani e agli italiani del Mezzogiorno. Faremo questa manifestazione per denunciare le vessazioni, le discriminazioni, il ricatto politico e la punizione politica che il centro‑sinistra ha stabilito per la Sicilia di Cuffaro così come per chiunque non abbia votato Prodi il 9 aprile. Il vice ministro D'Antoni e il vice ministro Capodicasa, qualche giorno fa, hanno impudicamente fatto il resoconto di quanta attenzione questo Governo ha dedicato alla Sicilia con la finanziaria. Avete deciso sgravi fiscali per i Comuni colpiti da fenomeni vulcanici, ma non è stato detto che le imposte in Sicilia si pagano alla Regione. Si fa festa a spese degli altri. Avete aumentato la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria di 1 miliardo e 112 milioni di euro in tre anni, ma ci si è ben guardati dal motivarla. Adesso aspettiamo il centro‑sinistra in quest'Aula per modificare questa norma. Avete deciso la cancellazione del finanziamento per il centro di biotecnologie Ri.Med, avete cancellato il ponte sullo Stretto di Messina. Vi state vendendo politicamente le risorse, che già erano della Sicilia e dei siciliani, come nuove risorse. Avete cancellato la più grande opera dell'ingegno umano, che avrebbe collegato direttamente all'Europa questo lembo di terra diviso dal mare Avete sottoposto lo Stato ad una causa di risarcimento danni con l'impresa vincitrice dell'appalto per un per un danno che farete pagare ai cittadini contribuenti. Avete detto che il porto di Augusta è un *hub* mediterraneo, ma questo è solo un riconoscimento di fatto che non tiene conto dei danni ambientali patiti a causa della raffinazione di petrolio che serve a l'Italia,

Miei cari amici del centro-sinistra, tutti possono sbagliare, ma meditate e ripensateci. Mi rivolgo soprattutto alla collega Finocchiaro, che sappiamo essere una spanna sopra la media della politica politicante.

prendiamo atto di tale volontà. Tuttavia, ci battiamo e continueremo a batterci affinché questa maggioranza possa cambiare idea e affinché quest'opera possa venire alla luce, visto che in cinque anni di Governo Berlusconi si era lavorato tanto, in maniera corretta e continua, affinché l'opera potesse venire realizzata.

questa richiesta non la sto rivolgendo certo a loro, ma soprattutto al Gruppo dell'Ulivo, la cui presidente senatrice Finocchiaro è certamente sensibile al tema che stiamo affrontando.

che la presidente Finocchiaro interverrà in proposito (la sollecito in tal senso), per consentire alla minoranza, visto il modo in cui si stanno conducendo i lavori, di poter dibattere più attentamente sui temi che residuano.

Presidente, spero che il senatore Ferrara si riterrà soddisfatto di come difenderò le ragioni del ponte. Ringrazio il mio Gruppo parlamentare per avermi lasciato questo spazio, avendo concentrato i minuti a disposizione per poter svolgere ragionamenti congrui e pertinenti su questa materia. Vorrei sottrarre questa materia, per la quale mi sono più volte battuto, alla polemica ideologica, per riportarla a contenuti di tipo economico. E per questa ragione vorrei leggere un intervento che ho scritto per tentare di convincere per l'ultima volta anche i colleghi

storicamente strategico per gli scambi commerciali tra l'Europa, i Paesi orientali, il Nord America e il Nord Africa. È un ruolo di grande piattaforma logistica, che ad oggi non può svolgere appieno per la mancanza di adeguate infrastrutture trasportistiche. La carenza e la inadeguatezza delle infrastrutture ferroviarie che collegano la Sicilia al continente portano ad una riduzione dei traffici, che prendono altre direttrici. Con la realizzazione del ponte, si eviterà completamente ogni possibile decadimento del livello di servizio e dei connessi fenomeni di congestione, grazie al marcato aumento della capacità del sistema di trasporto, e si potrà...

consentono il confronto nel merito. Sto tentando, cercando di abbassare i toni, di spiegare le ragioni per le quali non il Governo Berlusconi, ma un'intera classe dirigente, che ha attraversato legislature e responsabilità, ha considerato strategica quest'opera, ma quando finalmente quest'opera è stata avviata, è stata bloccata per ragioni incomprensibili. Questo è il dato politico, però vorrei ragionare su alcuni Lo Stretto rappresenta, inoltre, un ostacolo alla fluida circolazione di persone e beni: un collegamento stabile, aperto 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno è la migliore risposta alla domanda di un efficiente e moderno sistema di collegamento la Sicilia e il continente. Il ponte sullo Stretto consente di prolungare il sistema ad alta velocità e capacità ferroviaria nazionale ed europeo fino al centro del Mediterraneo. Infatti, l'alta capacità si ferma a Napoli e non raggiunge Reggio Calabria, perché il bacino di utenza calabrese non è sufficiente a dare una redditività, che invece si può ottenere aggiungendo i 5 milioni di abitanti della Sicilia, e l'attuale sistema di traghettamento non consente infatti il transito da e per l'isola di moderne tipologie di treni, come gli Eurostar, che possono essere utilizzati solo con un collegamento stabile qual è il ponte. L'opera non è stata progettata in maniera disgiunta dal contesto trasportistico locale e nazionale. Infatti, si colloca in modo funzionale ed organico in una logica complessiva di riqualificazione delle infrastrutture portanti del Mezzogiorno. Gli assi autostradali e ferroviari Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina saranno pronti in anticipo all'apertura al traffico del ponte, per la cui realizzazione sono previsti sei-sette anni di lavoro di costruzione, e il ponte rappresenta l'elemento trainante per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema dei trasporti meridionali. Ma il ponte, anche se rappresenta un'opera importante per l'inserimento della rete autostradale continentale in quella siciliana, è soprattutto determinante per lo sviluppo della rete ferroviaria a Sud di Napoli. Infatti, se si esaminano le tabelle allegate al mio scritto, che illustrano la flessione del traffico ferroviario merci e passeggeri attraverso lo Stretto, non si può non rilevare che la riduzione dei passeggeri è in netta controtendenza con lo sviluppo dei volumi di traffico nell'Italia continentale. È evidente che l'ostacolo costituito dalla necessità di traghettare i convogli ferroviari da Messina a Villa San Giovanni rappresenta un freno crescente allo sviluppo della modalità di trasporto ferroviario. Del resto, Ferrovie dello Stato, a fronte della costante riduzione della domanda, ha già più volte ipotizzato la soppressione del servizio di traghettamento dei convogli. Nell'ambito della strategia di rilancio degli assi portanti del Mezzogiorno, la realizzazione del ponte rappresenta quindi un efficace e determinante strumento di accelerazione. In tale prospettiva, non esiste alcuna contrapposizione tra il ponte sullo Stretto e le autostrade del mare ma, al contrario, c'è un forte rapporto sinergico. Solo con un collegamento stabile al continente gli scali portuali della piattaforma meridionale saranno altamente favoriti e competitivi con gli altri porti del Mediterraneo. Un sistema logistico più forte e competitivo si ottiene rafforzando le sinergie delle diverse modalità di trasporto, aria, terra e acqua, sviluppando così il concetto più volte ribadito di intermodalità. In assenza di un collegamento stabile, i porti siciliani saranno penalizzati rispetto a quelli direttamente collegati alla rete ferroviaria continentale. Un recente rapporto, commissionato da una primaria azienda di trasporti marittimi, mette chiaramente in luce i ritmi di crescita degli scambi commerciali, nonché le enormi ed uniche opportunità che ne possono derivare per l'area mediterranea. Nell'area occidentale e centrale del Mediterraneo fra il 2004 e il 2015 la domanda di movimentazione *container* crescerà del 75 per cento; i volumi fra il Mediterraneo e l'Estremo Oriente sono cresciuti nel 2003 del 19,4 e nel 2004 del 24,1 per cento e continueranno a crescere con tassi elevati. Analoga situazione si registra per gli scambi tra il Mediterraneo e il Nord America. Dunque, il Mediterraneo è una grande risorsa, ma al Mezzogiorno d'Italia e in particolare alla Sicilia non basta avere una posizione geografica strategica e solo con un efficiente sistema di rete ferroviaria il cui asse portante è l'asse ferroviario Palermo-Berlino, con lo snodo fondamentale del ponte, potrà avere un reale sviluppo economico e sociale. Per queste ragioni chiedo agli amici e colleghi che hanno sensibilità per i temi dello sviluppo del Mezzogiorno di superare gli schieramenti, di riappropriarsi di un'opera che è dell'intera classe politica di questo Paese se vuole uscire dalla congiuntura e guardare in termini di programmazione pluriennale, e votare a favore di questo emendamento per il quale chiedo il voto elettronico. Grazie

proposito del ponte sullo Stretto, una classe dirigente deve dimostrare di essere tale. Non è consentito al presidente Prodi di assumersi la responsabilità di dire che il ponte sullo Stretto bisognava farlo, quando era Presidente dell'IRI. Non è consentito ad una classe dirigente non ritenere che esista una continuità amministrativa. Non è possibile, per una classe dirigente che vuole qualificarsi tale, di

che ha deciso di volere fortemente la realizzazione del ponte sullo Stretto. Quindi, oggi non è possibile per questo Parlamento assumere un atteggiamento

deve dire sì alla realizzazione del ponte sullo Stretto, perché significa progresso, perché significa un ponte sull' Europa, perché significa la Sicilia al centro del Mediterraneo, creando condizioni di crescita per le giovani generazioni, per avere lavoro e prosperità, per avere un futuro degno di un futuro degno di una classe dirigente che sia garante del lavoro nella nostra terra di Sicilia. Non è dovuto alla politica chiedere di andare alla ricerca del lavoro, quando questo Governo dimostra ogni giorno di essere il Governo del no. No al ponte sullo Stretto, no ai termovalorizzatori, no a tutto quello che significa sviluppo per la terra di Sicilia. Ecco per quale motivo i senatori del centro-sinistra non hanno il coraggio di venire tra la gente di Sicilia, tra quella gente che ha detto sì alla realizzazione di questo grande progetto. Chiediamo,

anche alla luce dello storno dei fondi realizzati con questo decreto, nel senso della possibilità di realizzazione di quest'opera con altre risorse. Leggo l'ordine del giorno e chiedo ai colleghi la loro attenzione perché si tratta di un voto, ripeto, Presidente, su una affermazione di un principio, di un concetto, e quindi senza refluenza economica sulla tenuta del decreto: «Il Senato della Repubblica, in occasione dell'esame dell'articolo 2, commi 91-93, del disegno di legge n. 1132, considerati i trasferimenti delle risorse fino ad oggi stanziate per la realizzazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ad iniziative concernenti altri interventi infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in Calabria, impegna il Governo a ritenere non preclusivi i commi suddetti per la realizzazione del Ponte medesimo con altre risorse». Chiediamo, con questo ordine del giorno, se il principio della possibilità di realizzazione di quest'opera rimanga precluso o meno. Noi speriamo di no; possiamo avere chiarezza in quest'Aula da parte del Governo, riguardo al fatto che quest'opera possa essere realizzata o meno con risorse diverse da quelle stanziate nella società «Stretto di Messina»? Serve un'affermazione di coraggio:

che, una volta che si fosse votato l'emendamento di fatto soppressivo del trasferimento di fondi ad altre opere, si potesse dire che ciò non precludeva in via di principio

accelerare l'opera: si limita a dire (cosa peraltro molto importante) che il trasferimento delle risorse previste per il ponte ad altre opere da realizzare in Sicilia e in Calabria non è preclusivo del fatto che esso si possa realizzare con altre risorse. Quest'ordine del giorno non era stato distribuito prima; poteva essere presentato in Aula soltanto dopo la bocciatura del precedente

di questo decreto-legge, di non escludere che si possa egualmente dare vita all'opera. Come ha detto il collega Schifani, è una sorta di interpretazione autentica dei tre commi che prevedono il trasferimento delle risorse ad altre opere.

realizzare l'opera con altri fondi o se intende non realizzarla mai più. È un problema molto importante perché l'ordine del giorno è stato presentato in questo momento, signor Presidente. il collega D'Onofrio, che tra l'altro conosce bene la Sicilia, dove è stato anche amministratore locale, ha una grande speranza, quella che i colleghi della sinistra dicano: potremo farlo con altri fondi o in altra maniera. Evidentemente il collega D'Onofrio non ricorda le frasi di un ministro della Repubblica, Pecoraro Scanio, il quale ha affermato che non si farà mai più. Il presidente D'Onofrio dimentica quanto disse Rutelli in campagna elettorale; non parliamo di Prodi che lo disse tanti anni fa, ma può darsi anche che abbia avuto una mutazione genetica che lo ha portato ad avere altre sembianze da quando era Presidente della Commissione europea, presidente dell'IRI o grande *manager* di grandi affari. Rutelli in campagna elettorale ha detto: faremo il ponte. E poi, ha detto no al ponte.

votare), fu quello che quando uscì la tassa di soggiorno disse ai Comuni: ma perché questi inutili piagnistei, è una tassa da nulla, facciamola.

da presidente, ha firmato quest'ordine del giorno e noi siamo d'accordo: ma qui non abbiamo di fronte, lo dico all'amico Pistorio che tanto si è sforzato, un problema di tonnellate o di quintali. di un problema culturale e politico: bisogna far pagare alla Sicilia l'atteggiamento politico che la stessa ha, quando ha dato 61 deputati a 0 alla destra

Presidente, questa è la terza volta che devo intervenire sul modo in cui sia il relatore...

per la terza perché la votazione degli ordini del giorno ha luogo dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno espresso il loro parere.

che dice specificatamente: «Il Governo ed il relatore si pronunciano». Poiché in altre parti del Regolamento non è indicata la prerogativa del Governo con la parola «pronunciano»,

abbiamo visto che vi è una notevole sensibilità da parte della maggioranza su questo tema, il Governo non dia soddisfazione, non già soltanto ai componenti dell'opposizione, ma anche a quelli della maggioranza.

Presidente, mentre si svolgeva il dibattito relativo all'emendamento precedente,

è stato formulato e consegnato al tavolo della Presidenza e, immagino successivamente, a quello del relatore, soltanto in questo momento. Vorrei anzitutto confermare che nella Conferenza dei Capigruppo c'è stato un accordo politico, condiviso dal presidente Marini, per aprire un dibattito su tale vicenda e, successivamente ad un'eventuale bocciatura dell'emendamento, presentare questo ordine del giorno. Vorrei pertanto rassicurare non soltanto la minoranza, che anche oggi in qualche modo si è divisa su questa materia (è un aspetto che voglio sottolineare, perché secondo me è stato un errore),

sembra che da questa mattina abbiamo cercato in tutti i modi di venire incontro alle varie richieste, anche della maggioranza. non abbiamo concesso nulla e non vogliamo concedere nulla alla maggioranza. D'altra parte, la maggioranza da questo punto di vista però un dibattito senza interlocutori, perché abbiamo parlato solo noi.

alcuni aspetti di esso che sono fondati e lo sono a maggior ragione quando si arriva a scrivere un ordine del giorno all'ultimo momento, lo si presenta all'Aula,

più corretta ed efficace conoscenza del testo da parte dei colleghi. Ribadisco la celerità con cui il relatore, alzandosi, ha espresso parere negativo, richiamandosi ad un parere negativo su altro testo

lo ribadisco, si tende ad affermare un principio forte: l'opera può essere realizzata anche senza fondi statali o non deve essere realizzata in assoluto, anche in assenza di fondi statali?

Presidente, vorrei innanzitutto rassicurare i colleghi Cutrufo e Schifani che il relatore aveva ben compreso di quale ordine del giorno si trattasse e che lo stesso era stato distribuito già nella fase precedente l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

l'osservazione fatta dai colleghi in precedenza. In secondo luogo, quando mi sono apprestato ad esprimere il parere e lo stavo motivando, la signoria vostra, il Presidente,

abbiamo fatto la scelta qui in Aula, per ragioni afferenti all'economia dei lavori, di non ripetere argomenti già ampiamente svolti nella relazione, nelle repliche, in Commissione e in tutti i momenti nei quali sono stati discussi tali argomenti.

ed è questa la ragione per la quale confermo il parere contrario, cioè che i commi cui si riferisce l'ordine del giorno non sarebbero preclusivi alla realizzazione del ponte sullo Stretto. È una ovvietà: questi articoli non possono precludere alcunché; dispongono in termini positivi, nel senso che destinano le risorse per le finalità descritte nel decreto, ma non precludono alcunché. Se, invece, i presentatori vogliono discutere in quest'Aula in modo sostanziale se, quando e come sia possibile realizzare il ponte sullo Stretto, mi sembra che l'ordine del giorno ugualmente non possa essere accolto perché non affronta i problemi che una discussione di questo tipo richiede.

e promotore degli interessi del grande capitale finanziario, cioè delle banche. Basti pensare, per esempio,

italiana, a promuovere il blocco dello sviluppo della Sicilia ( poi andranno loro in Sicilia a spiegare il perché di questo impegno), perché volete fermarli?

E i senatori a vita, che vi sostengono, sostengono la minoranza elettorale di questa Camera. Questa è la vergogna di cui si coprono i senatori a vita

ad un intervento tale da poter far capire le volontà su un tema di grande prospettiva per l'Italia e per la Sicilia. Credo, allora, signor Presidente, che sia il caso di leggere...

Il ponte sullo Stretto...

Ritiro la mia firma dall'ordine del giorno e parlo in dissenso, non perché non sia d'accordo sul contenuto... PRESIDENTE. Mi scusi, lei è firmatario dell'ordine del

voglio ritirare la firma dall'ordine del giorno perché sono proponente di un emendamento, non di un ordine del giorno. È per questo che voglio motivare il mio dissenso e quindi il motivo per cui ritiro la firma. È chiaro? Non ho firmato l'ordine del giorno e c'è una ragione precisa, se possa esporla. PRESIDENTE. Ma lei non si deve inalberare perché le do io la parola in base al Regolamento, se lei non è chiaro io le chiedo perché parla. Quindi stia un attimo tranquillo, mi faccia spiegare.

Nonostante le dotte parole pronunciate ieri dal senatore Salvi e l'opinione del vice presidente Angius sull'equivalenza tra un emendamento e un ordine del giorno, c'è una profonda diversità di natura dell'atto; quella per la quale ho firmato un emendamento, ma non sottoscrivo e parlo in dissenso sull'ordine del giorno. Per la semplice ragione che l'emendamento, nel caso in cui venisse approvato, modifica la norma e quindi determina gli effetti di legge che vogliono essere raggiunti. L'ordine del giorno, anche qualora la maggioranza o il Governo lo accogliesse, o la maggioranza lo votasse, nulla ci lascia presagire che venga in qualche modo rispettato da questo Governo e da questa maggioranza. Abbiamo visto, infatti, anche in tempi recenti, mi riferisco per esempio, a ordini del giorno approvati durante la discussione del decreto Visco-Bersani, che il Governo non ha per nulla ottemperato. Per esempio, relativamente ad alcune fasi dell'implementazione dei sistemi di trasmissione telematica dei dati, posso portare un esempio recente per corroborare questa mia tesi, perché il Governo non solo è inadempiente rispetto al suo programma elettorale, cosa che avviene ormai con regolarità - perché la maggior parte, per esempio, delle norme che abbiamo in discussione su questo decreto fiscale non erano nel programma elettorale - ma è inadempiente anche rispetto alla sua maggioranza e a voti di questo Parlamento. Allora signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione

il suo tempo va nel contingente previsto per chi parla in dissenso. Quindi, quando sarà esaurito non potrà più parlare nessuno in dissenso. STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Concludo, perché non voglio sottrarre tempo ad altri colleghi che possono essere in dissenso. i colleghi, anche dell'opposizione, vogliono spiegazioni più dettagliate; posso anche impegnarmi in questo. Il punto chiave è il seguente: di fronte a progetti strategici per il Paese, di fronte a quello che era stato un progetto approvato dall'Unione Europea e cofinanziato, per ragioni puramente ideologiche e strumentali, la maggioranza ha deciso di stralciarlo e finge oggi di non voler sottrarre risorse alle Regioni meridionali, sostenendo che sono in qualche modo prioritarie altre opere. Prego i colleghi dell'opposizione di non prestarsi a questo gioco di propaganda per il quale anche l'eventuale approvazione del nostro ordine del giorno potrebbe fare il gioco di questo Governo inadempiente. Per queste ragioni, voterò in dissenso dal mio Gruppo.

non ci siamo espressi in nessuna maniera, quindi né con l'astensione, né con un voto a favore o contro sull'emendamento precedente. Useremo lo stesso atteggiamento

Non faremo nulla per il Brennero (che ci serve, serve agli altoatesini per andare in Baviera), non faremo nulla per il Frejus perché quattro scalmanati

essere sottoposti al ricatto perenne dei ricorsi al TAR che hanno sempre bloccato tutto. Riteniamo, quindi, in un'ottica federalista

dite no alle discariche, dite no ai termovalorizzatori, dite no al dragaggio dei porti, dite no alla BreBeMi che non costa una lira allo Stato italiano e che la voglion fare soltanto i lombardi. Dito no a tutto. State mandando in malora il Paese, questa è la verità! Pensateci! Altro che finanziaria di sviluppo! State fermando tutto! Non sapete nemmeno di cosa si parla, quando ci riferiamo alle aziende. Ma chi di voi è mai stato in un'azienda. Chi di voi, ditemelo? Nessuno di voi è mai stato in un'azienda!

mi sembra che la discussione si sia già sviluppata ampiamente. È stata data la parola a tutti i Gruppi e molti hanno parlato in dissenso e sull'ordine dei lavori. Credo sia il momento di passare alle votazioni. *(Alcuni senatori

un fatto di garbo, senatore Baccini. giorno G2.500, come spero possano fare tutti quei deputati siciliani che nelle interviste rese a Catania, a Palermo o a Messina si dichiarano a favore del ponte e poi qui assumono l'atteggiamento del silenzio o dell'ipocrisia, come fa il ministro Rutelli quando parla di turismo. Vorremmo anche sentire il presidente Ciampi, che in una visita a Messina dichiarò di essere...

ha dato la parola al relatore, premettendo che successivamente avrebbe fatto leggere al senatore segretario - queste sono le sue testuali parole - il testo dell'ordine del giorno. In ragione di questa sua affermazione e di una mancata distribuzione del testo, credo che molti senatori non abbiano contezza assoluta del contenuto dell'ordine del giorno. Le sarei grato,

senza ponte è evidente che la separazione creata dalla natura rimane, per cui bisogna votare per parti separate. Questa è la mia richiesta che non può essere superata come una semplice perdita di tempo. È un passaggio fondamentale previsto tassativamente dal Regolamento.

Presidente, su questo specifico argomento, perché un conto è votare per parti separate e un conto è capire quali sono le parti separate. Vorrei dunque venisse data lettura delle due parti separate su cui si deve votare.

Vorrei che l'Assemblea fosse messa a conoscenza di quali sono le parti separate, in modo che si possa votare

vostro è veramente un comportamento inaccettabile. Vi prego di fare attenzione alla lettura: è stato chiesto di leggere e pregherei di fare attenzione.

a ritenere non preclusivi i commi suddetti per la realizzazione del Ponte

votiamo l'ordine del giorno e quindi togliamo la seduta. Questa è una proposta della Presidenza. Se la proposta è accettata, possiamo procedere con i lavori, altrimenti continuiamo come stiamo facendo.

Colleghi, su questa proposta del senatore Malan, che è stata formalizzata, non c'è discussione, quindi chiedo all'Assemblea di esprimersi.

Presidente, si deve registrare un comportamento da parte di codesta Presidenza

Presidente. Il contingentamento dei tempi riguarda la discussione sull'Atto n. 1132. Se le chiedo Se le chiedo la parola, lei non sa per quale motivo la sto chiedendo; prima me la deve consentire, registrare la motivazione e poi, nel caso in cui la motivazione non sia ben posta, negarmi la parola. Lei per tre volte mi ha negato la parola. Il fatto che io l'abbia richiesta è certamente stato registrato nel resoconto e questo comportamento da parte di codesta Presidenza è di una gravità assoluta. PRESIDENTE. Grazie, senatore. devo parlare. Ora per allora, devo dirle che lei non mi ha consentito - ed è un mio diritto specifico - di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.500, cosa che certamente avrebbero voluto fare, differenziando il fatto che l'ordine del giorno riguardava per una parte Sicilia e per una parte la Calabria, i senatori siciliani.

parola e ho necessità che lei stia a sentire, perché le voglio ricordare che lei ha commesso un atto di una grande scorrettezza impedendomi di parlare Sì, cari colleghi, non c'entra niente, il gioco delle parti lo conosciamo: ho chiesto di parlare perché mi ero convinto della bontà dell'ordine del giorno e volevo aggiungere la mia firma *(Commenti

Non può ascoltarmi parlando con il senatore segretario. Le sto spiegando, caro Presidente, che lei mi ha impedito l'esercizio di un mio diritto.

che lei mi ha impedito di parlare: nonostante che il segretario dell'Aula, il collega segretario Viespoli, le avesse sottolineato che le chiedevo la parola, mi ha impedito di parlare. Allora, lei deve riconoscere che questo atteggiamento è assolutamente vessatorio. La ringrazio, signor Presidente. Diamo atto delle dichiarazioni del senatore Izzo, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno. Presidente, mi rivolgo a lei e le chiedo scusa per i toni con i quali prima mi sono rivolto alla Presidenza, però mi consentirà di considerare assolutamente inadeguata inadeguata la conduzione dell'Assemblea in quest'ultima ora. *(Applausi ironici Presidente Baccini, le ricordo che vige un Regolamento che anche il Presidente di turno è tenuto a rispettare e che quando le ho chiesto la parola, i funzionari, che fanno altri giochi, hanno fatto finta di non vedermi per evitare che lei... PRESIDENTE. Senatore Storace, la prego, si rivolga alla Presidenza perché i funzionari hanno fatto bene il loro lavoro. La prego di continuare. STORACE *(AN)*. Mi sto perché per Regolamento si ha il diritto di intervenire, di fronte ad una proposta del Presidente di Assemblea, per poter capire quali siano le parti che si intende far discutere, perché l'Assemblea ha diritto di conoscerlo. Poi lei ha ragione che si vota per alzata di mano senza discussione, ma il proponente ha il diritto di parlare, perché ha stabilito il presidente Marini, nonostante i funzionari, che questa è la regola in questa Assemblea. Lei ci ha impedito di poter rivolgere pacatamente argomentazioni perché dall'altra parte c'è stata una costante intimidazione nei confronti della Presidenza: lei ha avuto paura di essere imparziale, lei ha fatto sì che l'Assemblea fosse condizionata dalle grida dei nostri avversari politici. Questo è inaccettabile e la invito per il futuro a far rispettare anche questa coalizione.

*(FI)*. Signor Presidente, dobbiamo dare atto che è stata una seduta particolare, ci si è soffermato a lungo sulla trattazione di un argomento estremamente delicato. Io credo che, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, questa Presidenza sia stata sufficientemente attenta e paziente nel riconoscere il diritto alla parola all'Assemblea. Comprendo ed hanno tutta la mia solidarietà i colleghi che non hanno avuto la possibilità di intervenire perché ella ha ritenuto poi di procedere alle votazioni. In ogni caso, non potevo né intendevo astenermi dal fare queste considerazioni perché ritengo personalmente e politicamente che la conduzione dell'Assemblea di queste ore sia stata pluralista e democratica. Vorrei ricordare al presidente Schifani che la Presidenza non solo ha consentito di parlare a tutti i colleghi che lo volevano intervenire ma, in particolare, come ella sa, presidente Schifani, Forza Italia è andata molto oltre il tempo prestabilito e la Presidenza non ha fatto nulla per impedirlo.

Presidente, si è verificata una circostanza simpatica nel senso che la maggioranza sapeva che l'opposizione aveva a disposizione quattro ore di tempo per questo provvedimento

che anche i tempi per gli interventi sull'ordine dei lavori e per i richiami al Regolamento sono parte del contingentamento era evidente che i Gruppi che avevano esaurito i tempi non potevano più prendere la parola nemmeno sull'ordine dei lavori. Lei, Presidente, per un'ora ha dato la parola a tutti e mi stavo apprestando a dire che forse era un po' eccessiva la tolleranza della Presidenza.

comportamento che stavamo comprendendo perché anche noi ci facciamo carico delle esigenze della Presidenza di consentire la più ampia partecipazione. Abbiamo accettato questo confronto sul decreto fiscale ed anche compreso che l'opposizione, anziché quattro ore ne avesse otto. Presidente, penso veramente che sia stato un comportamento ingeneroso e anche la pezza che ha tentato di mettere l'autorevole Presidente del Gruppo Forza Italia,a nome di tutta l'opposizione, mi pare veramente un esempio di quelle iniziative che affondano ancora di più il coltello nella piaga. Vorrei, Presidente, dirle, con molta chiarezza, che a noi non è molto piaciuto che da quattro si sia passate ad otto ore; che a noi non è neanche molto piaciuto che, anziché concludere questa sera come era previsto nel tempo contingentato, si debba rinviare a domattina; non è nemmeno piaciuto - ripeto quanto detto stamattina - che l'opposizione sia stata un po' contraddittoria: da una parte, ha detto che si voleva un esame in Assemblea e che non vi era nessuna intenzione di forzare o di fare ostruzionismo perché si arrivasse alla fiducia; dall'altra, però si è comportata esattamente per arrivare a questo risultato. Ora, Presidente, in tutto questo bailamme, mi permetta di dire che noi ci auguriamo che domani mattina si possa riprendere i nostri lavori con il rispetto del Regolamento. Noi alla Presidenza dell'Assemblea chiediamo solo e soltanto questo: il rispetto del Regolamento. Poi comprendiamo le tolleranze, comprendiamo le disponibilità, comprendiamo tutto, ma, per piacere, quando c'è un'azione ostruzionistica come quella posta in essere dall'opposizione almeno il rispetto del Regolamento si impone per consentire a questa Assemblea di avere la sua dignità. *(Applausi ringrazio, senatore Boccia. Ribadisco e confermo che, indubbiamente, non solo il Regolamento è stato applicato, ma la Presidenza ha cercato di essere il più imparziale possibile e il tono degli interventi da una parte e dall'altra lo testimonia. Presidente, ho chiesto la parola non per lamentare il fatto che l'avessi ripetutamente richiesta e che lei non me l'ha concessa. Tenga presente che oggi ho svolto solo un brevissimo intervento per chiedere un chiarimento alla Presidenza in ordine alla proposta del senatore Malan di votare l'ordine del giorno per parti separate. Ho chiesto un chiarimento perché? Faccio questo intervento perché mediti su quanto è accaduto affinché non costituisca precedente per future occasioni. Il comma 5 dell'articolo 102 del «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione». Alla mia richiesta di specificare quali fossero le parti separate su cui si sarebbe dovuto votare, segretario ha letto l'ordine del giorno. Noi siamo stati costretti a votare senza avere nessuna specificazione su quali fossero le parti separate. Allora, delle due l'una: o non vi era stata alcuna specificazione e lei avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta di votazione per parti separate, ma - a mio avviso - non avrebbe potuto procedere alla votazione sulla proposta del senatore Malan, che non conteneva alcuna specificazione, né prima della mia richiesta, né dopo la stessa, sulle parti separate "Il link apre una nuova finestra"). Senatore Berselli, lei è troppo esperto per sfuggirle che il proponente, il senatore Malan, aveva specificato bene all'Aula, oltre che formalizzato successivamente, che le parti separate erano, da una parte, la Sicilia e, dall'altra, la Calabria. Poi, se vogliamo ovviamente andare oltre, ci potrebbero essere mille altre ragioni per puntualizzare. *(Il senatore Novi fa Presidente, le do atto che la sua gestione dell'Aula questa sera è stata ispirata al massimo della correttezza istituzionale, perché lei si è limitato ad applicare il Regolamento e, nello stesso tempo, non ha ha seguito gli indirizzi, anche verbali, provenienti dalla maggioranza parlamentare, che è minoranza elettorale. Il problema è il seguente. Vorrei ricordare ai colleghi del centro-sinistra, che hanno parlato di ostruzionismo, che quello di stasera non è ostruzionismo. Voi non sapete cos'è l'ostruzionismo parlamentare anche all'interno di questa Aula. Nella XIII legislatura, tra il 1996 e il 2001, l'ostruzionismo in questa Aula è stato tale da bloccare i lavori parlamentari, come ebbe anche a dichiarare il senatore Mancino, presidente del Senato in quella legislatura.

Voi qui non votate più nulla. Se noi vogliamo tutti quanti prendere la parola sul Regolamento, voi qui non votate più nulla.

verso il ruolo dell'opposizione. Infatti basta leggere i resoconti del Senato - la mancanza di rispetto esternata dall'allora opposizione nei confronti della Presidenza Pera, le aggressioni anche fisiche nei confronti della Presidenza Pera i tentativi di delegittimazione nei confronti della Presidenza Pera - per rendersi conto che questa opposizione, che è maggioranza elettorale, nei confronti della Presidenza e del Governo ha sviluppato

la minoranza elettorale a tener conto della situazione all'interno di quest'Aula. È intollerabile il costituirsi di una sorta di partito oligarchico dei senatori a vita. Non è mai avvenuto nella storia del Paese che i senatori a vita esprimessero omogeneamente il sostegno ad un Governo. Si fa riferimento a quanto avvenuto nel 1994; allora però i senatori a vita, sulla

furioso lo è stato nella legislatura precedente, come frusta nell'altro ramo del Parlamento; dimentico lo diventa oggi quando afferma che in dissenso non si potrebbe intervenire o quando fa riferimento al contingentamento. La sostanza del mio intervento, però, è un'altra: non accetto che un senatore autorevole della maggioranza possa dire che non gli è piaciuto ciò che è avvenuto in Aula: Aula: è un senatore della maggioranza, non un giudice del nostro comportamento. A questo punto, però, mutuo il suo modo di parlare e dico che a me non piace il fatto che a lui non sia piaciuto, perché ciò non deve avvenire, nel senso che il suo non può essere un giudizio di merito sui comportamenti; può essere, di converso, un comportamento politico sui comportamenti che abbiamo tenuto. Le dirò di più.

Sono andato dal senatore Boccia e gli ho detto: «A questo punto, procediamo domani con le dichiarazioni di voto». Lo stesso senatore Boccia ha risposto che questo non poteva essere fatto, con ciò negando un accordo raggiunto precedentemente. A questo punto, è nato quello che può essere giudicato

la possibilità della posizione della questione di fiducia e poi avrebbe consustanziato questa realtà. Il nostro comportamento è conseguenza di una condotta

se fosse stato accolto il suo invito, così come aveva chiaramente detto, di rinviare la discussione, dopo quella votazione, alla giornata di domani, forse la tensione si sarebbe certamente stemperata. Dobbiamo darle atto di avere accordato ogni possibilità di espressione anche del dissenso; quindi non c'è stata nessuna compressione e questo è un elemento di garanzia per quanto riguarda l'andamento dei lavori parlamentari. Colgo anche l'occasione, Presidente, per rinnovare ancora una volta l'invito affinché nella giornata di domani la Presidenza del Senato possa farsi interprete affinché sia presente il Ministro dell'economia e delle finanze o il vice Ministro. Se questo decreto fa parte della manovra finanziaria, ciò richiede tale partecipazione soprattutto nelle fase finali, altrimenti ci sarebbe una sottovalutazione del ruolo del questo Senato.

proprio per evitare di parlare, come dire, a Senato pieno, con il rischio di una strumentalizzazione delle riflessioni che, invece, pacatamente vorrei fare sul piano politico e istituzionale rispetto all'andamento dei lavori. Vorrei dire al senatore Boccia che la dialettica parlamentare è tale quando il Parlamento è sovrano nelle scelte, quando cioè - e lei me lo può insegnare attraverso il dibattito, il confronto, il Parlamento ha la possibilità di cambiare, di votare e quando la maggioranza o la minoranza hanno la possibilità di individuare punti di convergenza comuni su un provvedimento. La dialettica parlamentare è tale quando può decidere, non quando può ascoltare e fare testimonianza di posizione politica. Voi avete impostato questo decreto con una sorta di fiducia mascherata,

attraverso i giornali e nelle sue esternazioni televisive, aveva addirittura chiesto che sugli ordini del giorno ci fosse la copertura finanziaria. Io non avevo colto questo elemento, come dire, innovativo, fortemente innovativo. Ascoltando il dibattito, ho capito perché il ministro Padoa-Schioppa aveva chiesto che addirittura sugli ordini del giorno ci fosse la copertura finanziaria: perché la dialettica parlamentare è consistita fin dall'inizio - addirittura attraverso le parole del Presidente della Commissione Bilancio

del determineremo, del cambieremo. La maggioranza, senatore Boccia, era consapevole sin dall'inizio della blindatura del provvedimento relegando il ruolo dell'opposizione alla testimonianza e non

attraverso la blindatura della maggioranza. Questa, infatti, ha determinato ordini del giorno per cui sull'ICI e sulla tassa di scopo sostiene

proviene dal Garante dell'unità nazionale. Il Capo dello Stato, garante dell'unità azionale, individua un senatore a vita per pregi, per qualità, perché ha onorato la Nazione nel campo della cultura, della scienza, dell'arte. Poi, vi sono i senatori Presidenti emeriti che, per definizione sono stati custodi dell'unità nazionale.

Chiarezza istituzionale significa che, probabilmente, basterebbe cambiare una norma del Regolamento. Basterebbe stabilire che i senatori a vita, a meno che non scelgano diversamente in termini di appartenenza ai Gruppi, non fanno parte del Gruppo Misto, ma di un Gruppo diverso.

perché il senatore a vita, se la fonte della sua legittimazione è quella, non può trasferire la propria rappresentanza. Io sono stato eletto in una lista e io posso trasferire ad un altro senatore del mio Gruppo e del mio partito la presenza nella Commissione. Il senatore a vita è stato scelto *intuitu* *personae* e non può delegare la presenza in Commissione. Basterebbe questo a chiarire, dal punto di vista della dignità delle istituzioni e del Senato,

adesso, arrivato al Senato e ritrovatosi nella maggioranza, fosse anche lui affetto da celiachia politica, cioè da intolleranza alla critica e all'opposizione.